L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

su una questione che le illustro brevemente. Come sa, domani noi avremmo calendarizzato il disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito con la clausola «ove concluso», ma il citato provvedimento non arriverà in Aula, Aula, nonostante ci sia stato un impegno a calendarizzarlo per l'Assemblea in settembre. Tra l'altro, la richiesta delle opposizioni era che il disegno di legge fosse calendarizzato prima della pausa estiva, ma non si è potuta ottenere questa calendarizzazione. Ricordo che si tratta di un disegno di legge

che dobbiamo esaminare perché la Corte costituzionale in più occasioni ha chiesto al Parlamento di legiferare in materia. Tuttavia, la ragione per la quale il disegno di legge non arriverà in Aula è che quando siamo stati

Tanto per dare l'idea, noi siamo riuniti adesso alle ore 16 di lunedì, in via abbastanza straordinaria, mentre le Commissioni 2a e 10a si sono riunite alle ore 14,45 di oggi perché ci sono tutte queste audizioni da fare.

commercializzazione della *cannabis* *light*, alle sanzioni ai detenuti che protestano in modo non violento, all'occupazione delle case. Si tratta, insomma, di un disegno di legge di grandissima complessità complessità e, quando abbiamo chiesto un numero congruo di audizioni, ci è stato detto da un esponente autorevole della maggioranza che si trattava di una manovra ostruzionistica da parte delle opposizioni.

devo fare cento audizioni di cento associazioni che dicono tutte la stessa cosa, cioè non c'è alcun approfondimento in termini di maggiore conoscenza per il legislatore che si accinge a legiferare, non abbiamo alcun valore aggiunto; quando, invece, andiamo a trattare argomenti distantissimi gli uni dagli altri, tutti inseriti all'interno di uno stesso disegno di legge, che, tra l'altro, signora Presidente, non è calendarizzato, quindi noi non abbiamo alcuna

che la Presidenza del Senato mi aiutasse a comprendere un punto: se le audizioni servono ad approfondire materie complesse e delicate, come il fine vita, ne dobbiamo fare cento, allora, quando parliamo di restringere i diritti e le libertà dei cittadini con un provvedimento così invasivo, io mi aspetto di poterne fare altrettante. Soprattutto non mi aspetto di sentirmi dare dell'ostruzionista appunto, sempre col mio cappello di senatore della 2a Commissione, sto facendo audizioni addirittura il lunedì pomeriggio o alle 8 di mattina, perché ne dobbiamo fare la richiesta sull'ordine dei lavori era di un chiarimento su quale debba essere anche l'utilizzo da parte delle Presidenze delle Commissioni di questo strumento così utile come l'audizione, perché non possiamo fare che quando le audizioni le chiede la maggioranza possono essere date a centinaia, quando le audizioni vengono chieste dall'opposizione bisogna mettersi d'accordo con dei numeri risicati.

Senatore Scalfarotto, ferma restando l'autonomia delle Commissioni di stabilire l'ordine dei propri lavori, lei sa che questo tema è già stato affrontato in Conferenza dei Capigruppo, ma certamente può essere approfondito in quella sede.

quando analizziamo i decreti e presentiamo gli emendamenti, nel senso che ci siamo accorti strada facendo che, rispetto a quella che era negli ultimi tempi una procedura di individuazione, ovviamente rispetto a quello che prevede il Regolamento, di quelli che sono considerati gli emendamenti estranei per materia, quindi non ammissibili al testo del provvedimento; noi eravamo abituati - almeno io ricordo - nella vecchia legislatura al passaggio che c'era

di recente notiamo con sempre maggiore frequenza che c'è anche un ulteriore parere, diciamo così, di ammissibilità che arriva da istituzioni superiori. Quindi, vorremmo capire la procedura chiedendo che magari lei, Presidente, si possa far carico di comprendere bene questo passaggio, in modo tale che noi ci sappiamo regolare, perché se noi sapessimo prima quali sono gli emendamenti che possono essere più o meno considerati ammissibili a un testo, allora saremmo orientati, nelle prerogative del Parlamento, a segnalare quelli che sono considerati ammissibili, in modo tale che ci possa essere una discussione e un confronto più sereno. Segnalare prima alcuni emendamenti considerati prioritari dai Gruppi per poi dopo sentirci dire che alcuni non vanno bene, perché, ripeto, ci sono delle legittime istituzioni che possono intervenire e fare delle valutazioni, pone un problema di procedura che mi piacerebbe approfondire, magari in un'apposita Conferenza dei Capigruppo, ferme restando sempre quelle che sono le prerogative esclusive

esclusiva dei Presidenti di Commissione. Tutte le altre interlocuzioni avvengono nel rispetto del Regolamento, oggi così come ieri. Certamente si può approfondire anche questo tema nella Conferenza dei Capigruppo. Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"

al Paese. Sono intervenuti diversi emendamenti, anche al di là di quelli presentati come relatore, insieme al collega Lotito. Mi fa piacere che ci sia stato un coinvolgimento totale di tutte le forze politiche. È un provvedimento che abbraccia più aree, più settori del nostro Governo, del nostro Stato,

tutti quei provvedimenti di proroga che possono aiutare, soprattutto nell'ambito degli enti locali, l'attività di sviluppo e di crescita del nostro Paese. Un'attenzione dimostrata soprattutto dalle approvazioni che ci sono state e soprattutto un lavoro di sintesi importante che è stato fatto su un argomento specifico, quello degli enti locali, dove siamo riusciti, anche grazie al contributo da parte delle opposizioni, a far sì che si potessero approvare degli degli emendamenti importanti e fondamentali, per far sì che anche i piccoli Comuni potessero ritenersi sollevati rispetto a delle incombenze di carattere burocratico. gli emendamenti importanti che posso citare, uno è quello relativo alla facilità dell'entrata in servizio dei segretari comunali, in modo tale da garantire, anche ai piccoli Comuni, di fare più velocemente e di essere più attrattivi rispetto a queste figure professionali, professionali, importantissime e fondamentali per l'attività degli enti locali stessi. Si è intervenuti nell'ambito fiscale. Siamo intervenuti con un importante emendamento, che è quello relativo al concordato preventivo biennale, che sicuramente, al di là di quelle che sono le dichiarazioni che ho letto sugli organi di stampa in questi giorni, probabilmente deve essere spiegato meglio.

ringrazio i Commissari per la disponibilità che hanno dimostrato, in termini di orario e di presenza, anche nei giorni festivi. Questa è una dimostrazione di attenzione verso l'Italia, verso la crescita del nostro Paese, che noi, attraverso l'approvazione di provvedimenti come quello di oggi tendiamo a portare avanti.

Presidente, dopo la relazione esaustiva fatta dal mio collega, Giorgio Salvitti, c'è poco da dire. Vi sono alcuni temi fondamentali che sono stati affrontati e che rappresentano sicuramente delle novità. Mi riferisco alla lotta alla pirateria, che sicuramente porterà dei ricavi importanti e soprattutto debellerà un'azione in mano alla criminalità organizzata, che oggi gestisce questa attività. Soprattutto, determinerà il rispetto di quelli che sono i valori sia della società, ma soprattutto i valori delle azioni che vengono messe in campo per debellare questo fenomeno. Noi abbiamo emanato una norma, che purtroppo poi ha avuto scarsa applicazione, per delle criticità che sono emerse. Noi abbiamo inteso, d'accordo con l'Agcom e d'accordo con le autorità preposte, di andare a rimuovere queste criticità. Lo abbiamo fatto con una norma che, attraverso un emendamento, risolve tecnicamente tutti i problemi. Abbiamo puntato la nostra attenzione soprattutto su alcune iniziative di carattere fiscale che sono fondamentali per rimettere in moto l'economia e dare certezza del diritto a coloro che, dal punto di vista formale, si sono trovati

di risolvere il problema del termovalorizzatore e della criticità idrica che attanaglia la Regione Sicilia. Insomma, abbiamo adottato una serie di iniziative - lo ripeto - in un clima di grande collaborazione anche con le opposizioni (che hanno dimostrato grande senso di responsabilità),

in modo indefesso: lo dico perché tutta la giornata di domenica l'abbiamo trascorsa a cercare delle mediazioni su alcuni punti che poi sono state trovate; tali mediazioni hanno consentito di redigere un testo che porterà dei grandi risultati, contrariamente a quello che qualcuno vuole

un lavoro puntuale e soprattutto condiviso, all'insegna delle mediazioni e del risultato pratico.

Signor Presidente, certo che a sentire le affermazioni dei relatori mi viene un po' da sorridere; anche loro hanno sorriso guardandoci e c'è un motivo. Mi riferisco al fatto che noi abbiamo una visione totalmente diversa rispetto a questo provvedimento che oggi discutiamo in Aula: forse nelle intenzioni avrebbe dovuto essere veramente un atto finalizzato a decidere importanti misure a favore dei cittadini; ahimè, è solo una scatola vuota o, meglio, un calderone in cui trovano spazio misure che poco incideranno sulla vita delle persone e soprattutto delle imprese. Per far crescere il Paese servono misure strutturali, una visione, una politica industriale che guardi al medio e lungo termine. Oggi, invece, siamo di fronte e ci troviamo a votare

del Governo che io stessa ancora non ho ben capito: abbiamo capito che hanno stanziato 100 milioni di euro per dare 100 euro a determinate categorie di lavoratori, ma chi è la veramente la platea di questi beneficiari? tanti paletti e tante condizionalità che rendono veramente impossibile capire la norma: fino a quando ero solo io a non capirla poco male, se non fosse che anche il Vice Ministro, venuto in audizione, ha dichiarato che ci saranno

In realtà, caro Vice Ministro e cari colleghi della maggioranza, quei bambini hanno bisogno di tutto, dalle scarpe ai vestiti e un accesso alla scuola sereno però il Vice Ministro ci dice che ci saranno dei correttivi, come fa sempre questo Governo, in ogni atto che porta in Commissione e in Aula. Ormai vi abbiamo conosciuto, infatti: voi siete quelli del "poi"

del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che è al 18 per cento dello stato d'avanzamento della spesa del PNRR e, ancora, del PNC. E noi cosa facciamo? Togliamo quelle risorse che servono allo sviluppo del Sud per accontentare e far far bello un Ministro - che ormai fu Ministro, visto che sta andando a Bruxelles - che aveva individuato soltanto 1,8 miliardi per una ZES unica del Mezzogiorno, che è impossibile coprire solo con tale importo. La ZES unica al Mezzogiorno non serve, perché abbiamo tolto le specialità, ma soprattutto senza senza un piano infrastrutturale non abbiamo risolto il problema del Sud. Il Sud - e lo dice una che viene dal profondo Sud - non ha bisogno di piccoli incentivi, ma di certezze e questa ZES stanzia somme soltanto per un anno, il 2024. Ma un'impresa investe investe solo se ha l'incentivo per un anno? Occorre almeno per un triennio, perché bisogna parlare a lungo raggio con le imprese, dando certezza delle azioni.

all'inaugurazione della Fiera del Levante a Bari, ho sentito la Meloni dire che quest'anno il Sud è stato la locomotiva economica dell'Italia, a differenza degli anni passati: nel 2023 il PIL del Sud è cresciuto più della media nazionale, l'occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al resto d'Italia e gli investimenti sono cresciuti del 50 Presidente, ma che affermazione è? Solo propaganda mistificatrice della realtà, che non è neanche vera, perché basta andare a vedere negli anni passati: già agli inizi degli anni '80 e nella metà degli anni '90, il tasso di crescita del prodotto interno lordo per abitante nel Mezzogiorno d'Italia aveva superato il corrispondente tasso di crescita nazionale circa un anno su tre. Lo stesso è accaduto nel medesimo lasso di tempo al tasso di crescita del prodotto interno lordo per abitante nelle isole. Lo stesso è accaduto fra la metà degli anni '90 e i primi della decade in corso, e la Meloni non c'era. Quindi non è l'azione che sta facendo questo Governo che porta ogni tanto questo PIL *(Applausi)* ad alzarsi nel Mezzogiorno, ma sono i piani

senza sottrarle ad altri programmi - e, soprattutto, di una politica con un approccio meno democristiano dello sviluppo da Cassa del Mezzogiorno. Non vogliamo più sentire quella parola. Vogliamo una politica industriale di attrazione di investimenti, anche per cambiare il paradigma. Non voglio più sentir dire "resto

Noi siamo ad esso contrari nel merito, come ho detto in Commissione, e soprattutto perché, come già hanno dimostrato le associazioni ambientalistiche che hanno presentato un ricorso, non c'è attualmente alcuno stato di emergenza inerente alla gestione dei rifiuti in Sicilia. un disperato bisogno di guardare agli affari che conseguono alla costruzione degli inceneritori, che cancelleranno ogni progresso ottenuto nel perseguire la raccolta differenziata. Una raccolta difficile in Sicilia, dopo dieci anni di Governo di centrodestra. Ricordo infatti che le percentuali di raccolta differenziata

Stando così le cose, non può che trovarci del tutto contrari soprattutto la nomina di un commissario straordinario senza il requisito della straordinarietà e la reale scadenza del mandato e soprattutto senza i limiti imposti dalla legge del codice degli appalti. Le deroghe non riguardano il diritto europeo dei contratti pubblici e neppure le misure antimafia; questo ha dichiarato Renato Schifani ieri alla stampa locale in Sicilia. Per placare le polemiche dice che serve soltanto per tagliare i tempi di alcuni passaggi amministrativi e accelerare la fase di progettazione. Presidente, così però ci troviamo di fronte allo stravolgimento della Costituzione perché, come ho detto in Commissione, il presidente Schifani ha dei problemi ad affrontare il dibattito pubblico. I termovalorizzatori per essere inseriti in un piano stralcio ed essere approvati, così come prevede la norma sul codice degli appalti, deve prevedere un dibattito pubblico. Lo stravolgimento della Costituzione e la concentrazione di poteri nelle mani di una sola persona, uniti alla totale discrezionalità sulla durata dell'incarico, fanno di Schifani non solo il presidente della Regione, ma un viceré. Manca la cerimonia di incoronazione, ma i poteri sono i medesimi. Trovo la crisi istituzionale nel quale questo Governo sta precipitando la Patria ancora più complessa e profonda se inquadriamo questa nuova figura di viceré di Sicilia nella più ampia strategia di demolizione delle istituzioni democratiche che questo Governo sta perseguendo. Il Governo Meloni continua con l'occupazione delle posizioni di potere della Nazione, lo stravolgimento della Costituzione, il cambiamento della forma di governo in Italia con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'annullamento di fatto del bicameralismo e delle funzioni del Parlamento. Per quanto mi riguarda, fino a che mi consentono di esplicitare le mie funzioni di parlamentare, voglio ricordare a tutti noi - se la storia può insegnarci qualcosa - che quando Roma, tra le tra le cui rovine viviamo oggi, concentrò troppo potere e denaro nelle mani dei pochi, la Repubblica venne cancellata per dare spazio agli imperatori.

dei numeri macroeconomici per gli anni in corso e, quindi, anche per gli anni futuri. In certi casi stiamo parlando di questioni sostanziali che poi magari vedremo. In realtà, dentro questo decreto-legge ci sono alcune cose che erano il poi del passato. Faccio un esempio tipico. Ripeto: stiamo parlando di manutenzione e non stiamo risolvendo i problemi del mondo, ma i problemi di qualche categoria. Una di queste categorie è quella di chi,

in Italia (campeggi, per intenderci, così almeno sappiamo di cosa parliamo) è molto rilevante e la contribuzione al PIL vale esattamente quanto quella dell'esportazione di un manufatto di alta tecnologia che in certi casi ci lascia stupefatti e ci fa dire quanto siamo bravi e quanto è brava la nostra industria. Dal punto di vista dei conti dello Stato, un banale campeggio in realtà contribuisce alla nostra crescita esattamente nello stesso modo, perché significa soldi da parte di stranieri che arrivano nella nostra economia, aiutandoci ad avere più agio e più possibilità di spendere anche per questioni molto importanti quali le detassazioni, gli incentivi e i rinnovi dei contratti. Se non hai contratti. Se non hai un incasso da una parte, difficilmente, con le regole attuali, potrai avere una spesa dall'altra parte (anche la più importante, come quella per la sanità). Non è mai una cosa staccata da un'altra. In tre Governi della scorsa legislatura ho sempre provato a far passare la norma di minimo buonsenso che chiarisse che una casa mobile è mobile. Sembra strano farlo capire, ma in realtà, a quanto pare, il concetto che una casa mobile sia mobile non passava all'interno della macchina dello Stato perché

con nessun tipo di omogeneità all'interno dello Stato (dipendeva dalla fortuna del luogo dove il campeggio era dislocato), diceva che non importa che ci sono le ruote, ma che interessava lo scarico. E se per caso c'era uno scarico, allora doveva pagare l'IMU. Da lì venivano fuori dei contenziosi assolutamente assurdi che poi, ovviamente, si concludevano con la ragione del povero campeggiatore. Tuttavia, capite bene che quella che doveva iniziare come una pacifica attività imprenditoriale (o, peggio ancora, una vacanza) diventava un incubo. Finalmente, dopo tanti "poi" e dopo tante situazioni (Governo Conte I, Governo Conte II e Governo Draghi) in cui questa cosa non era mai riuscita a essere sistemata, adesso è andata a posto, con grande soddisfazione degli operatori del settore. Piccole cose? Sì, piccole cose.

Se delle eccellenze di maestri di musica arrivano in Italia per studiare, questo va anche al di là dell'introito del singolo maestro. Ciò significa uno strumento di promozione e di e di lustro dell'Italia nel mondo, perché, quando questo maestro andrà a esibirsi nei teatri e nelle orchestre di tutto il mondo, nel suo *curriculum* ci sarà, come

Era la proroga di un finanziamento per il 2027 e, quindi, non è un poi, ma è un guardare un po' avanti. È evidente che accademie di questo livello devono avere la possibilità di programmare i lavori e non possono pensare di iniziare adesso un'attività didattica che poi finisce nelle nebbie. Ringrazio tutti i colleghi che hanno supportato questa idea

come modello per quello che vogliamo fare in futuro. Io penso che ci sarebbero meno litigiosità in quest'Aula e, dall'altra parte, più soddisfazione da parte dei cittadini, perché si troverebbero uno scenario un po' più sgombro da certe pastoie burocratiche eredità di un lontano passato. In certi casi si vanno a sanare questioni che veramente risulta incredibile pensare da quanto tempo sono state strutturate. Queste cose sono visibili - e questa è, se possibile, un'attività di cui il Parlamento deve essere fiero - grazie all'attività dei parlamentari sul territorio, perché non sempre è possibile rendersi conto che qualcosa non quadra.

cerchiamo, per quanto possibile, di capire che i vagli di ammissibilità non hanno con sé soltanto un aspetto che che inerisce alla soddisfazione del singolo parlamentare che ha faticato, che ha pensato di mettere giù un emendamento, ma spesso e volentieri hanno dietro delle storie che magari potrebbero avere un consenso unanime. Cerchiamo di rendere tale procedura la più trasparente possibile. Dietro ogni emendamento scartato, ci sono numerose richieste e delusioni da parte di chi invece vorrebbe, magari a buon diritto, trovare sanata una situazione analoga a analoga a quelle che prima ho delineato e che siamo riusciti a sanare. Invece, purtroppo, la pallina non ha girato dalla parte giusta della roulette e quindi non ha funzionato. Un minimo di rispetto per tutti gli emendamenti presentati dalla maggioranza e dall'opposizione deve essere - secondo me - la nostra bussola per il lavoro futuro. Questo è stato un caso particolare, perché c'era pochissimo tempo per lavorare. Per i decreti futuri, mi auguro che ci sarà più tempo per valutare quanto c'è di buono nelle proposte dei singoli parlamentari.

registro con favore l'intervento del senatore Borghi Claudio, che, a differenza dei toni utilizzati da altri colleghi della maggioranza, ha definito questo provvedimento un decreto di manutenzione. Io lo definirei un decreto di manutenzione pasticciato, con interventi a volte anche inutili e dannosi; lo specchio fedele di una politica economica senza prospettiva, senza

Il testo originario vede un credito di imposta per gli interventi del Mezzogiorno ancora non adeguatamente finanziato; vede misure di carattere economico con impatto sull'attuazione del Piano nazionale complementare, a cui però sono state sottratte risorse, nonché norme su società a controllo pubblico, sul sistema di istruzione, formazione e ricerca, su attività culturali, sugli investimenti nel Continente africano e sugli enti territoriali. Insomma, la sostanza evidenzia un provvedimento non solo pasticciato - come dicevo prima - ma anche inutile, perché non risolve e neppure mette in una prospettiva di risoluzione tutta una serie di nodi, a conferma della poca cultura riformatrice del Governo. Il quadro, se è possibile, è stato ulteriormente peggiorato in Commissione tra tempi contingentati, mancata collaborazione del MEF sui pareri agli emendamenti e mediazioni dentro la maggioranza avvenute tutte in sede extraparlamentare. La prima versione per l'accesso al concordato preventivo per gli evasori senza sanzioni, con il pagamento di una tassazione simbolica per gli anni di imposta 2013-2018, era un vero e proprio schiaffo ai contribuenti onesti. Anche la versione definitiva, dopo le svariate proteste, non muta la sostanza, l'idea che anche gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale. Il concordato preventivo, tramite lo strumento del ravvedimento, è un pessimo messaggio verso tutti quelli che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco. Riflessioni a parte meritano due pacchetti di norme: quelle sulla giustizia e quelle sul *bonus* Natale, che si iscrivono pienamente nella deriva ideologica che il Governo ha imboccato su queste materie. Sulla giustizia - proprio nelle settimane in cui, con il decreto sicurezza, si introducono 20 nuove misure tra inasprimento delle pene e nuove fattispecie di reato, seguendo in questo la logica di un populismo penale inefficace ai fini della sicurezza - si finge di mostrare il volto feroce come nel caso dei gestori del servizio di accesso alla rete per omessa segnalazione di IP pirata. Ma poi questo giustizialismo a buon mercato si scioglie come neve al sole quando, dall'altra parte, non c'è un capro espiatorio da dare in pasto all'opinione pubblica per palesarsi come insofferenza alle regole. Insofferenza alle regole è quella che si ritrova nella totale deroga alle norme del codice degli appalti per il commissario rifiuti della Sicilia, a cui viene conferita tale facoltà anche per interventi riguardanti la siccità, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica. È quella che continua sul fronte delle regole urbanistiche e catastali delle procedure edilizie: si assiste a disposizioni come il superamento catastale degli allestimenti mobili nei campeggi, alle regole della doppia conformità per taluni manufatti. Unica nota positiva del provvedimento sono alcune disposizioni sul fronte degli enti territoriali che, grazie all'iniziativa dell'opposizione e agli emendamenti depositati, hanno risolto alcune delle problematiche del comparto. Il massimo, però, lo si raggiunge con il *bonus* Natale, misura manifesto per la prossima campagna elettorale, che invece riguarderà una platea ristrettissima di persone, escludendo dal beneficio i contribuenti con figli nati fuori dal matrimonio: una vera e propria discriminazione di Stato costruita da un Governo che crea bambini di serie A e di serie B per rincorrere e alimentare la loro farisaica idea di famiglia. E allora, Presidente, questo Governo si accinge a scrivere la sua terza manovra e la canzone resta sempre la stessa: non ci sono risorse, dobbiamo tenere in ordine i conti pubblici. Ma la verità è che, dietro questi obiettivi che - vale la pena ricordare - hanno riguardato tutti i Governi degli ultimi trent'anni, si cela un vuoto di idee senza precedenti su come dare spinta e competitività alle nostre imprese; su come fare in modo che lo sviluppo economico cammini di pari passo con la transizione ecologica; su come costruire un sistema più equo e più giusto sia dal punto di vista fiscale, sia da quello del rafforzamento della concorrenza del libero mercato. Nulla di tutto questo si è visto fino ad ora. Nulla di tutto questo si trova nel decreto-legge in esame, che invece ben fotografa i vizi e i limiti di questo Governo nelle materie fiscali e della crescita economica. Diminuiscono i soldi e si tagliano i servizi a partire dalla sanità. Ma, nel frattempo, il debito comincerà a scendere solo dal 2027, e non per garantire la coesione sociale e i diritti delle persone, ma solo per garantire gli interessi innanzitutto di elusori ed evasori;

ossificando per sempre disparità non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centri urbani e aree interne. Signora Presidente, come Partito Democratico ci opporremo con forza a questo

di carattere fiscale e ordinatorio ed è anche legato a incentivi importanti in termini di economia e di sviluppo dei territori; basti pensare alle misure sulla zona

a cercare di dare una copertura importante in termini di risorse a quegli imprenditori che realmente vogliono investire e non vogliono aspettare semplicemente la manna dal cielo.

Ci sono misure fiscali nel campo dello sport che, in un'ottica di semplificazione, prorogano le agevolazioni IVA delle associazioni sportive dilettantistiche e che apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l'erogazione di corsi e attività sportive invernali, per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri Paesi.

Per i 220 nuclei familiari destinatari dei provvedimenti di sgombero per inagibilità dopo il crollo, il Governo ha previsto un contributo mensile fino a che non troveranno una sistemazione stabile e comunque entro la fine dell'anno 2025. Una somma aggiuntiva è prevista anche per le famiglie con persone anziane e disabili.

Sono stati stanziati ben 13 milioni di euro a sostegno del turismo dei Comuni situati all'interno dei comprensori delle aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze turistiche causata dalla mancanza di precipitazioni nevose nel periodo dal novembre 2023 al marzo 2024. Le risorse saranno destinate alle imprese turistiche operanti nei Comuni dei comprensori delle aree sciistiche della dorsale appenninica che, nell'arco di tempo preso in considerazione, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 Con questo intervento ribadiamo ancora una volta il nostro impegno a sostegno della montagna italiana, che si conferma *asset* strategico per il comparto anche nel periodo estivo, tanto da far segnare un aumento delle presenze rispetto a quelle dell'anno scorso. Il Governo sta dalla parte delle imprese che contribuiscono fortemente a trainare l'economia nazionale. Sono previste anche misure di chiarimento per il versamento di imposte a favore di enti locali e l'applicazione della legge della *spending review* per quanto riguarda le Regioni. C'è il tanto vituperato *bonus* Natale,

la norma non è chiara. Ebbene, il sottosegretario Leo - ho assistito alla audizione - ha precisato i contorni di questa norma, che derivano anche dalla necessità di inquadrarsi in un articolo ben preciso del Testo unico sui tributi e, quindi, ha delle caratteristiche dovute a questo. Chiaramente, come per tutti i provvedimenti di origine fiscale, poi saranno pubblicate delle circolari di applicazione che serviranno a spiegare meglio l'ambito di azione. Poi c'è il famoso emendamento che è stato approvato, relativamente ai poteri commissariali della Regione Sicilia, per quanto riguarda i termovalorizzatori. e di fatto che cos'è questa norma? È una norma che dà al presidente regolarmente eletto della Regione siciliana, il Governatore, quei poteri che ha il sindaco di Roma, ad esempio, che servono ad accelerare - sì - un processo importante, che è quello della realizzazione dei termovalorizzatori in una realtà che sicuramente deve fare molto e sta facendo in questo contesto per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ma poi esiste comunque una una grande produzione di residuo indifferenziato, che in questo momento mandiamo all'estero, e lo mandiamo in Danimarca, dove evidentemente - la verde Danimarca - i termovalorizzatori funzionano. che vogliamo fare? Realizzare dei termovalorizzatori in Sicilia, in aree già individuate, con un percorso nell'ambito della legalità e nel rispetto di tutte le norme nel tempo più veloce possibile. Questa norma non fa altro

Non stravolge assolutamente il contrasto alle infiltrazioni mafiose. E sarà fatta seguendo tutti i protocolli di massima attenzione da questo punto di vista, anche con l'ausilio della Guardia di finanza. Sta seguendo un percorso importante, perché il piano rifiuti sta sta passando nella Commissione di merito della Regione siciliana, ed è stato inviato anche al Consiglio di giustizia amministrativa, che in Sicilia è l'organo superiore della giustizia amministrativa per il controllo preventivo. Chiaramente c'era un percorso che prevedeva altre lungaggini amministrative che, con questa norma, vengono ridotte. Quindi, non si vuole stravolgere nulla, non si vuole creare alcuna dittatura, ma si vuole semplicemente dare una risposta ai cittadini siciliani e - vivaddio - è compito di qualsiasi Parlamento e di qualsiasi Governo. Altre norme sono state approvate riguardanti gli enti locali e i segretari generali dei Comuni. Grazie all'apporto dell'opposizione sono stati approvati altri emendamenti, esempio sul bonus psicologo, su cui evidentemente c'è stato un lavoro importante. Ringrazio i colleghi della Commissione e i relatori che, anche nei giorni festivi, hanno lavorato alacremente a questo provvedimento, che - come tutti i provvedimenti di urgenza - chiaramente sconta la necessità di comprimere i termini e i tempi del dibattito parlamentare, e non perché si voglia - come sempre viene invocato - costruire un regime in cui la democrazia parlamentare viene negata, ma semplicemente perché si vuole cercare di intervenire nel più breve tempo possibile per le necessità che hanno i nostri cittadini. Vedete, in una società nella quale oramai la velocità di comunicazione e di azione si misura in secondi, probabilmente alcune norme nascono già vecchie quando vengono pensate e, quindi, molto spesso dobbiamo intervenire con la procedura d'urgenza, che non è quella classica parlamentare, quella principale di approvazione

di eccezionalità e sicuramente riguardano tanti aspetti della vita della nostra comunità nazionale che attenzioniamo nel nostro agire quotidiano. Noi abbiamo superato il secondo anno di Governo Meloni. ma i sondaggi continuano a dare il massimo della credibilità alla *Premier* Meloni e alla coalizione che la sostiene, confermati - se mi consentite - dai risultati delle elezioni europee e delle varie elezioni regionali che si sono susseguite. a volte non viene percepito immediatamente, perché è un lavoro duro, umile, determinato, che consiste anche di provvedimenti come questo, che non hanno norme eccezionali da raccontare. Sono, però, provvedimenti importanti, che riguardano la vita delle persone. Rappresentano la cifra di un Governo che è improntato al realismo, alla sana attenzione agli equilibri della finanza pubblica e, nel contempo, ad utilizzare al meglio le risorse che noi abbiamo a disposizione per investimenti che abbiano un senso reale e una reale capacità di di migliorare quel sistema amministrativo, anche negli enti locali, sul quale tanto noi ci spendiamo e al quale noi tanto crediamo. Quindi, un provvedimento su cui convintamente noi voteremo a favore. È un provvedimento provvedimento importante e, onestamente, tutto il resto sono discussioni che non interessano ai cittadini italiani. Signor Presidente, Governo, senatrici e senatori, mi perdonerete se non mi soffermerò sul provvedimento tutto nella sua interezza. Lo abbiamo avversato e lo diranno e lo hanno detto assai meglio di me i colleghi che hanno lavorato in Commissione, che ringrazio, che ne hanno maggiore competenza e contezza. Non parlerò, insomma, dell'ennesimo condono, dei quali si è perso ormai il conto: dai contanti, alle tasse concordate, al salvacalcio. Ieri, in Commissione, sempre sul pallone, siamo stati paralizzati per ore su uno su un dissidio all'interno della maggioranza, tra il coriaceo senatore Lotito e gli affannati Capigruppo della destra, accorsi, meschini, di domenica a placare le ire del presidente, lo Stakanov dell'emendamento, il Torquemada del "pezzotto", il tormento di Garavaglia, l'incubo di Calandrini. Dicevo dei condoni della destra: uno al mese, forse di più, dallo stralcio delle cartelle agli scontrini, agli scudi penali, alla rottamazione *quater*, alle multe, le criptovalute, gli avvisi bonari, la conciliazione agevolata, concordati, sanatorie, rateazioni, la tregua fiscale per arrivare alla pace edilizia; tutto ciò con questa neolingua che ieri arrivava a definire il solito "condoncino" un ravvedimento operoso, neanche il senatore Orsomarso, con tutto il rispetto, fosse un gesuita del Seicento: non è perdono, senatore,

una vita meno esangue. Hanno l'illusione, per pochi minuti e per pochi spiccioli, di contare qualcosa, addirittura di esistere o, come nel caso dell'opposizione, di resistere. Un formaggio fatto di subemendamenti, accordicchi, telefonate convulse, manfrine, piagnistei, misirizzi, piazzate: uno spettacolo d'arte varia, al quale ormai sono ridotti e confinati la nostra

siamo riusciti tutti insieme - vorrei sottolinearlo - a portare a casa due milioni di euro in più sul *bonus* psicologo per l'anno in corso. *(Applausi)*. Ne avevamo chiesti 25 per il 2024 e 50 per il 2025, dal momento che, delle oltre 400.000 richieste arrivate all'INPS negli scorsi mesi, soltanto poco più di 3.000 più di 3.000 potranno accedere a questo sostegno: meno dell'1 per cento. Come sapete, il *bonus* è nato all'indomani della pandemia, quando l'ombra della salute mentale ha rivelato a poco a poco la sua estensione e il suo impatto, la sua violenza nella vita di ognuno di noi e in particolare delle generazioni più giovani: una epifania di fragilità, di friabilità, che non avevamo saputo cogliere, presi dall'emergenza delle vite da salvare, del respiro che mancava, dell'incubo di quelle settimane e di quei mesi di Covid-19. Altro che uno per cento, signor Presidente! Nel Lazio credo siano poco più di un centinaio le persone ammesse ad avere questo piccolo sostegno economico per affrontare un percorso terapeutico. È per una misura che invece funziona, che ha dimostrato di funzionare e di essere apprezzata da tutti: da chi ha bisogno di un aiuto, dai terapisti, dalle famiglie. Non nascondiamoci, allora, dietro la scarsa dotazione per dire che questo sostegno non serve: serve eccome e va finanziato adeguatamente. Ieri abbiamo messo due milioni sul 2024. ma il prossimo anno si riparte da otto milioni. Erano 25 all'inizio: siamo andati molto indietro e ogni volta ci ritroviamo all'ultimo secondo, strappando quel che si può alla Ragioneria generale, ai Ministeri, e poi si vedrà. Ma non può funzionare così. Il *bonus* va inserito all'interno di un'offerta adeguata sulla salute mentale da parte dello Stato. Lo psicologo di base nelle scuole e negli atenei non può e non deve essere un pannicello caldo, un alibi, una pezza da mettere a tutto ciò che manca. Sulla sanità, colleghi, manca moltissimo, direi manca quasi tutto. Figurarsi sulla salute mentale, che arriva sempre dopo tutto. Cito inoltre i tumori, gli infarti, il pronto soccorso. Presidente, le vorrei dire che ci sono tante perplessità sul ricorso ai *bonus* per il loro carattere temporaneo, emergenziale. Il Governo ha digrignato i denti - basta *bonus* - salvo poi proporne uno natalizio. Evidentemente ci sono *bonus* e *bonus*: se sono miei, sono più *bonus*; se non sono miei, sono meno *bonus*, magari dimenticandoci che queste misure dovrebbero essere non nostre o vostre, ma per tutti. Non è che io non condivida le resistenze sui *bonus*, l'ambizione che ciò che resta che si faccia strutturale, come questa misura, peraltro, che ha ormai carattere permanente. C'è un "a decorrere" lì, e quindi, è uscita ormai dalla evanescenza delle misure aspettando la grande riforma e gli investimenti massicci per la salute che finora non si è stati proprio in grado non dico di assicurare, ma neanche di immaginare (e quando avete avuto l'occasione, con la proposta del Partito Democratico, l'avete lasciata cadere); aspettando la grande riforma doverosa, sacrosanta ed epocale, intanto le persone stanno male. Lo Qualche giorno fa, signor Presidente, il neo nominato *premier* francese Barnier di un Governo di destra ha indicato come priorità per la sua azione quella della salute mentale. In Gran Bretagna il neo *premier* Keir Starmer, che la presidente Meloni ha conosciuto e - mi pare - apprezzato, nonostante la diversa collocazione politica, ha indicato nel "discorso del re", tra i punti qualificanti del suo programma di legislatura, la salute mentale. E così avviene negli Stati Uniti, in Germania e in Europa. Non si tratta, insomma, di destra e di sinistra, ma si tratta di noi, Presidente, e lo dico al Governo. Ieri, se non avessimo trovato la sponda dell'Esecutivo e della maggioranza che ha sottoscritto il nostro emendamento, sarebbe passato in cavalleria e di questo vi va reso onore. Signor Presidente, io però non ci dormo la notte a pensare che, per 3.000 persone che avranno un incentivo, ne restano 370.000 che sono rimaste fuori e che magari avevano e hanno molto bisogno, necessità e urgenza. Io non ci dormo la notte per i ragazzi che si tagliano le braccia e le gambe in cameretta. Io non ci dormo la notte per i tentativi di suicidio, per la solitudine nel chiasso dei *social*: isole che, come tutte le isole, anelano a naufragare o sprofondare. Non ci dormo la notte per i corpi sbriciolati, il ciclo che non viene, i denti che cadono; per il cibo come veleno, per i farmaci buttati giù come acqua. Non ci dormo la notte per i pianti delle madri, per il baratro dove ti ritrovi senza accorgertene; per la corsa alle strutture di assistenza e di ospitalità che ci sono, ma che sono poche e che hanno quei posti lì. Non ci dormo la notte alle fughe, alle bugie, alle telefonate notturne, alla vulnerabilità estrema, alla violenza sofferta La salute mentale è un allarme nazionale e globale: riguarda le vite di ognuno di noi, delle persone più care, di chi amiamo, dei nostri amici, dei nostri figli, di noi stessi, occhi aperti al buio. Non possiamo andare avanti mangiucchiando qualche milioncino qua e là: dobbiamo prendere sul serio le persone che non ce la fanno. Quanto a quelle che invece grazie a un percorso terapeutico oggi sono fuori: una mia amica, qualche giorno fa, mi ha mandato le foto della figlia, dopo un calvario di anni, in spiaggia con altri ragazzi felici. *(Applausi)*. Oggi, con questa posta minima, 1.300 persone in più potranno iniziare il loro percorso per ritrovarsi: non sono niente, sono 1.300 persone. Di questo però non dobbiamo essere orgogliosi, colleghi, ma sentirci responsabili per tutti coloro che resteranno inascoltati, che non hanno i soldi per provarci, che non sanno dove sbattere la testa, che stanno pensando di farla finita. So che nessuno di noi in quest'Aula farà finta di niente. Ci sono priorità ed emergenze, lo so, ma questa riguarda davvero ciascuno di noi, la nostra ombra, come quella dello Schlemihl di Chamisso, dalla quale non possiamo separarci, pena perderci. Abbiamo adesso davanti manovre di bilancio, milleproroghe e altri provvedimenti. Noi ci riproveremo ogni volta, ma solo insieme, come quando si perde la strada, se ne esce solo insieme. *(Applausi)*.

intanto, prima di esaminare il testo in esame, vorrei ricordare che ieri, nella giornata di domenica, abbiamo celebrato la Giornata mondiale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. di un evento che non può passare in sordina perché è importante: evitare lo spreco alimentare, soprattutto oggi, è un modo per sostenere l'economia delle famiglie, ma anche l'ambiente. La lotta allo spreco alimentare rientra nei piani dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

e prevediamo addirittura la possibilità di ordinare porzioni ridotte (le cosiddette miniporzioni), allo scopo di ridurre al massimo la quantità di cibo prodotta non consumata, a beneficio soprattutto del consumatore stesso e della sostenibilità dell'ambiente.

di interesse sono molti: segno della costante attenzione del Governo a sostegno delle varie categorie, dell'economia e del Paese. Si interviene per adeguare una serie di norme alle mutate necessità della società e dell'economia in uno scenario difficile, che purtroppo non accenna a mutare; anzi, vediamo che ogni giorno si complica sempre di più. Esso segna la continuità dell'azione che hanno già portato

forte e la possibilità di accedere a un ravvedimento speciale per gli anni 2018 e 2022 per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale. C'è anche una serie di agevolazioni molto più veloci per di ripresa e resilienza. È vero: questo emendamento prevede anche più tempo per i controlli per le partite IVA che non aderiscono al ravvedimento nei termini di decadenza dell'accertamento che erano al 31 dicembre 2024 e sono stati prorogati al 2025; per quelle che aderiscono sono invece prorogati al 31 dicembre 2027. Tali interventi potrebbero servire da traino allo stesso concordato. Fondamentale è l'emendamento che semplifica il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione che mira ad assicurare a tutti gli attori della filiera attuativa la liquidità necessaria per realizzare gli interventi prevede che i trasferimenti successivi all'anticipazione siano erogati dalle amministrazioni centrali titolari delle misure entro trenta giorni dall'acquisizione delle richieste di erogazione. Segnalo poi una misura importante a sostegno delle famiglie, che introduce il *bonus* di Natale di 100 euro per le famiglie con figli fino a 28.000 euro di reddito. Si tratta di un'indennità esentasse da erogare con la tredicesima e che vale per 1,1 milioni di lavoratori per cento dei lavoratori dipendenti), per una spesa complessiva di circa 100 milioni di euro. Vi sono poi anche gli emendamenti approvati per debellare la pirateria *streaming*, pure per gli eventi sportivi:

l'altro obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete che vengono a conoscenza di condotte penalmente rilevanti di segnalarle immediatamente all'autorità o alla polizia giudiziarie. Positivo è il contributo straordinario da 10 milioni di euro:

C'è anche una risposta chiara ed esaustiva ai piccoli Comuni che hanno un grave problema di carenza di copertura di posti dei segretari comunali. Sono state introdotte nuove regole per ridurre i tempi per l'immissione in servizio di nuovi segretari comunali, con l'obiettivo di superare la storica carenza di iscritti nella fascia iniziale di accesso a questa carriera. Un emendamento dà la possibilità

Un emendamento a firma del nostro Gruppo propone il termine di differimento per l'IVA al 5 per cento sulle cessioni dei cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Secondo il testo attuale, l'aliquota ridotta si applica entro i diciotto mesi dalla nascita: con l'entrata in vigore di questo emendamento - che non è banale - il nuovo margine temporale sulla vita del puledro, che si conteggia per l'aliquota ridotta, diventa il 31 dicembre dell'anno successivo. Diamo una risposta concreta a un'esigenza che da anni il settore ci chiede.

a delle scelte nei cui confronti questo Parlamento è così lontano, soprattutto nel rendere gli emendamenti fattibili di discussione e di approvazione. Certo è che mi auguro che quest'Aula e le Commissioni competenti possano prendere in esame

e alcuni dei risultati - in realtà assai pochi rispetto a quelli cui ambivamo - che sono stati raggiunti nei lavori della Commissione. Nell'approssimarsi dei due anni dall'elezione di una nuova maggioranza nelle Camere, che il provvedimento al nostro esame, il primo con il quale siamo partiti dopo l'estate, nella mia esperienza di membro della Commissione bilancio, è stato il più raffazzonato, il più mal gestito come tempi, il più incerto nel dialogo con il Governo. E ciò è tanto vero che, alla fine, moltissimi emendamenti non hanno potuto trovare neanche un'analisi da parte del Governo.

è stata veramente la peggiore alla quale abbiamo assistito. Spero che sia un effetto estivo e non invece un nuovo corso dopo i due anni, e cioè stabilizzazione dell'approccio di questo Governo. Pensate che noi abbiamo iniziato i lavori il 4 settembre e ancora ieri, domenica, ci siamo riuniti per capire quali tipi di emendamenti potevano essere accolti. Devo ringraziare tutte le forze politiche, permettetemi di partire da quelle di opposizione, che hanno insistito fino alla fine per porre il tema del grande capitolo degli enti locali dentro questo decreto *omnibus*. Noi abbiamo insistito moltissimo. Abbiamo tenuto la barra dritta e, grazie a questo e al confronto con i parlamentari della maggioranza, alcune piccole misure sono state ottenute. È poco però: noi avevamo centinaia di emendamenti segnalati dall'ANCI, per esempio, e da Comuni che hanno tantissimi problemi di stabilizzazione. Noi dovremmo cercare

problemi nell'assunzione, nel reperire personale e nel fare delle proroghe. Tutto questo va sistematizzato e ci vuole un intervento *ad hoc*. Naturalmente, accanto alle cose positive - poche - che siamo riusciti a fare (è stato citato prima il *bonus* psicologo,

La prima riguarda la ZES. Noi abbiamo criticato la ZES tante volte e vi abbiamo spiegato che occorreva una ZES differenziata, cioè una misura per distinguere, all'interno del Sud, le aree Sud, le aree che hanno più bisogno di sostegno, altrimenti tutte le misure finiscono per andare sempre negli stessi posti. Vi dicevamo che la copertura che avete previsto è insufficiente. Questa cosa oggi avviene e ci viene data ragione. Ma cosa si fa? Si usano risorse del fondo complementare del PNRR per finanziare e cercare di dare maggiori risorse alla

8 euro al mese che diamo soltanto a chi riesce ad avere tutti i requisiti, ossia, sostanzialmente, ai coniugati con figli a carico. a carico. Mi chiedo perché dobbiamo escludere alcune famiglie. Mi vengono in mente tante donne, tante ragazze madri che sono sole, che sono italiane, che sono cristiane, che sono delle mamme e magari hanno anche dei nomi diversi da quello di Giorgia e un reddito inferiore ai 28.000 euro. Perché questo modello di famiglia non vi piace al punto tale da eliminare qualunque tipo di incentivo per queste madri? All'interno dei 28.000 euro c'è inoltre una distribuzione completamente diversa. Qui stiamo spendendo 100 milioni per anticipare, prima delle elezioni regionali, una misura sulla quale siamo pronti a discutere perché ha degli aspetti positivi: mi riferisco alla defiscalizzazione e detassazione delle delle tredicesime. Tuttavia, anticiparla con i vincoli che sono stati detti significa semplicemente prendere 100 milioni e buttarli in un contesto nel quale non dovete pensare che 8 euro al mese possano moltiplicare la domanda e, quindi, far crescere il PIL in Italia.

che non risolverà alcun problema, ma creerà inequità e disparità e alimenterà le disuguaglianze, lasciando fuori tantissime persone che effettivamente avrebbero bisogno. Quanto al condono, non è che se continuiamo a chiamarlo

Questo non era il Governo della deterrenza, che è partito con il *rave party*? Non è un Governo che crede che norme più dure disincentivano le persone dal commettere reati? Se credete questo, allora dovete anche dire alle persone che evadono o non pagano le tasse che non avranno alcun trattamento di deterrenza. Voi state incentivando il ritardo nel pagamento delle tasse. Quindi, sostanzialmente, state rendendo strutturale un messaggio di questo Governo cui chiunque debba pagare delle tasse può sempre farlo in ritardo, perché alla fine ci sarà la possibilità di aggiustare le cose. Questo porta molte meno entrate di quelle di cui il Paese ha bisogno.

al commissario di Roma, che in realtà ha un altro tipo di copertura legislativa. Si fa una confusione estrema, perché sostanzialmente si semplifica moltissimo e si tolgono delle responsabilità che sono anche del precedente governatore Musumeci, e alla fine si mettono insieme rifiuti e acqua, per quanto la norma parli soltanto di rifiuti. Una grande confusione, in una Regione martoriata dall'incapacità di gestire la questione dei rifiuti e dall'incapacità di contrastare le infiltrazioni mafiose in quel settore. Alla fine ci sono due norme. La prima cancella una norma dell'Antitrust, che l'Antitrust stessa ha detto essere anti-concorrenziale; non si comprende il motivo di questa norma. L'altra è quella che ha citato il collega Lotito, che non vedo in Aula. Per il suo tramite, Presidente, gli vorrei dire che non esiste al mondo una norma di questo genere, che dice che, se qualcuno è a conoscenza di qualcun altro che sa che qualcuno sta facendo pirateria, e non interviene, si fa un anno di carcere. Questa cosa non c'è in nessuna parte del mondo. Capisco che poi alla fine bisogna trovare degli equilibri, ma questa è una norma che non regge un minuto nel contesto europeo. Qual è la qualità legislativa che si produce con questi decreti decreti *omnibus*, se poi alla fine si negozia qualcosa non - come ha detto un collega che mi ha preceduto - che chi è a conoscenza lo segnala, perché la norma non dice questo. La norma dice: se non lo segnali, ti fai un anno di reclusione. È scritta talmente male che venire a conoscenza non sappiamo che cosa significhi; sono questioni di cui si deve occupare l'autorità. Concludo, Presidente, dicendo che tutto questo, finita l'estate e a inizio dei lavori parlamentari, ci dà un'altra idea. Qui non si sta facendo la storia o perlomeno, se si sta facendo la storia, la si sta facendo nel modo peggiore: la storia da dimenticare e non da imitare. È una storia rispetto alla quale, a due anni dall'inizio della legislatura, anche gli italiani si stanno rendendo conto che non è, come si dice da altre parti, una storia infinita da ripetere, ma una storia da chiudere al più presto, per il bene delle italiane e degli italiani.

Devo dire che non si vede una grande omogeneità: infatti è *omnibus* perché c'è un po' di tutto al suo interno. Riprendo la domanda che ha fatto il collega capogruppo Romeo e che io, modestamente, ho posto domenica in Commissione:

un altro emendamento, che era stato completamente dimenticato rispetto all'*omnibus* iniziale. forse dovremmo capirci. Nessuno ha presentato oggi una questione pregiudiziale di costituzionalità, perché penso che ci sia anche una certa stanchezza nel presentarla inutilmente. Però una risposta dal Presidente del Senato dobbiamo averla; dobbiamo averla; se un decreto è *omnibus*, le inammissibilità dovrebbero essere considerate forse con minor rigore. È stata fatta già una preselezione, infatti poi, subito dopo, i Presidenti hanno chiesto alla maggioranza di sfoltire gli emendamenti

di Inter e Milan: siamo sicuri che i presidenti di calcio siano così sensibili alla necessità di stroncare la criminalità organizzata? Da quello che si legge in queste ore, mi pare di no, ma capisco che invece sui diritti televisivi c'è un interesse economico importante e quindi quella norma ha una priorità, per gli interessi personali del presidente Lotito, molto più forte rispetto ad altri interessi. Quello che mi ha veramente fatto sorridere è che tutte le misure, quelle sì, di manutenzione inerenti alla vita vera sono state respinte. Una su tutte quella sull'assicurazione per i trattori nelle strade: quanti trattori vanno in strada e quante falciatrici vanno in strada? Penso

quello che viene indicato come l'emendamento che dà potere al presidente Schifani di ovviare alle norme del codice degli appalti: questa manutenzione mi interessa, perché quando fu approvato il codice degli appalti di salviniana memoria, si disse che lo si faceva per abbreviare abbreviare tutto ciò che era ordinario e finalmente i commissari che, fino a quel momento venivano nominati per velocizzare le procedure, sarebbero scomparsi così, con un battito di ali. E invece no, prevedete un commissario. A parte che la prima versione della norma era completamente sbagliata e ve ne siete accorti cammin facendo, perché per cercare di dargli un po' di onorabilità si legava il commissariamento degli impianti al PNRR, poi qualcuno ha detto che gli impianti del PNRR non comprendono i termovalorizzatori, ma tutto quello che riguarda l'economia circolare, perché la parola "termovalorizzatore" è stata espunta all'epoca in cui fu approvato il PNRR. Allora avete cancellato il riferimento

però: nell'emendamento che avete individuato non fate le gare, date un affidamento *in house* alla municipalizzata della Sicilia che - devo dire dubito che brilli per efficienza, perché altrimenti non avrebbe bisogno del commissario Schifani, ma ci arriverebbe da sola a fare il termovalorizzatore. *(Applausi)*. Quindi, se si vuole accelerare ed efficientare il sistema dei rifiuti siciliano, forse la gara, la gara, quella vera, aperta anche ai privati, con tutte le garanzie del caso e i controlli di sicurezza per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata, andrebbe fatta. Noi abbiamo visto veramente gli emendamenti più disparati, che non hanno nessun collegamento, e lo dico in mente quello che è stato chiamato il *bonus* Befana. Chi vi parla è sempre stata orgogliosa del *bonus* di 80 euro del Governo Renzi, che poi è stato massacrato nel corso dell'opera e adesso non ha più quella visione. Quel *bonus* aveva un senso innanzitutto perché non era un *bonus*, ma un taglio al costo del lavoro e perché andava alle persone. alle persone, senza trattino, senza dover fare una classifica. In questo caso, invece, avendo 100 milioni e dovendo dare un contentino, si è fatta una classifica una classifica che il vice ministro Leo ha cercato di spiegare e più la spiegava e più io mi sono detta: poveri imprenditori che dovranno dare questo *bonus.*

ma non hanno diritto di essere scambiate per evasori. Hanno l'obbligo di avere diritti - questo sì -, di avere delle garanzie - questo sì - e non di essere considerate

ma un modo per rendere simpatico un Governo che non sta dando risposte alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori italiani. eccomi qua, sono ricomparsa; richiamate tutte le unità,

siete riposati, siete stati con le vostre famiglie, avete ricaricato le batterie, molto bene. Ha detto addirittura: siete persone fortunate, perché potete fare questo in questo Paese. Secondo me, però, non avete contezza di quello che sta succedendo veramente in questo Paese, fuori da quest'Aula. La situazione è drammatica:

ci sono stati 2.070 fallimenti per problemi di difficoltà finanziaria; 11.000 sono le liquidazioni volontarie. Avete completamente affossato il PIL, la crescita è immobile in questo Paese, il lavoro si è sviluppato, ma è un lavoro povero. che farete buon uso e trarrete energia da quello che avete messo da parte in questo periodo estivo e avete concluso dicendo che siete pronti.

Non so cosa sia successo, ma da quando è arrivato settembre le sedute d'Aula sono sempre di meno e le Commissioni saltano di continuo. Non so se sono state troppo lunghe queste ferie, oppure se i treni purtroppo non funzionano bene non riuscite a arrivare a Roma, o siete troppo presi dalla vostra tele-Meloni che racconta di tutto tranne quello che succede nel Paese, dalle questioni di Boccia

Il decreto-legge di cui parliamo oggi è stato licenziato il 9 agosto e siete dovuti correre in emergenza domenica 29 settembre per non farlo decadere. Secondo me, non avete capito come funziona, oppure è stato troppo il tempo perso da questa Commissione e dall'Aula. L'Assemblea che non sta lavorando da due settimane. Lavoriamo pochissimo, le sedute di Commissione sono sempre più ridotte: questo è lo specchio di quello che non state vedendo. Questo è lo specchio di quello che non capite e che succede fuori da quest'Aula. Questa è la dimostrazione che siete completamente lontani dalla realtà e raccontate quello che volete raccontare a televisioni unite, come pensate di risolvere i problemi, ma non si risolvono così i problemi. C'è una questione in particolare - questo decreto

c'è un tema che ricade fortemente in questo decreto, fra i tanti che avete inserito, che è quello dell'azzardo. L'azzardopatia è un problema di questo Paese e quindi avete inserito in questo decreto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professioniste, società e associazioni sportive dilettantistiche. Allora ci può andare bene, ci può anche stare che lo Stato conceda un credito d'imposta, un'agevolazione fiscale a qualcuno che non pagherà imposte, perché investe in pubblicità.

maniera subdola, il gioco d'azzardo, come sono tutti quei siti di *infotainment* che girano in rete e che riempiono i campi da calcio in questo momento. è stato bocciato, non c'è stata neanche la possibilità di affrontare una discussione. Lo sapete quanto fatturano queste aziende nel nostro Paese? Paese? Nel 2019 queste aziende hanno raccolto nel nostro Paese 110 miliardi che arrivano da cittadini, persone in difficoltà, famiglie che spesso e volentieri sono quelle maggiormente in difficoltà, che buttano i soldi in questo tentativo di cambiare il loro futuro.

Purtroppo, il periodo della pandemia ha rialzato i dati relativi alla questione del gioco, che è ricaduta di nuovo sulle famiglie fragili, sulle persone in difficoltà, così nel 2021 siamo ritornati a 111 miliardi e nel 2022 a 136 miliardi.

Come la Sottosegretaria ha annunciato, nel libro blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 2023 siamo arrivati a una raccolta di 149 miliardi, che arrivano tutti quanti dalle famiglie italiane, dalle famiglie italiane, tutti quanti dalle tasche delle famiglie italiane: 149 miliardi. E noi, a fronte di una raccolta del fisco che va da poco più di 12 a 15 miliardi, a queste aziende diamo un credito d'imposta. A me sembra surreale quello che sta succedendo.

perché sia chiara e rimanga agli atti di questa discussione. Sapete quanti sono gli italiani che hanno dei problemi di azzardopatia in questo Paese? Lo chiedo ai patrioti. Lo sapete quanti italiani si rovinano la vita? Un milione e mezzo di italiani si rovina la vita: loro, le loro famiglie, tutte le persone che hanno intorno, tutti i loro amici e tutti quelli che hanno a cuore queste persone. Sono un milione e mezzo. *(Applausi)*. Solamente per dare dei dati e capire quanti sono i tossicodipendenti in questo Paese, rispetto ai dati

Coloro che si rovinano la vita, il proprio futuro e quello della propria famiglia e dei propri figli con l'azzardopatia, sono un milione e mezzo di italiani e noi diamo loro la possibilità di raggiungere le informazioni in maniera ancora più diretta, in maniera ancora più concreta; non solo questo, ma agevoliamo anche

Però, ci terrei a sottolineare un altro di questi temi, che è drammatico. Questo decreto lo ha fatto venire fuori ed è importante che se ne parli in quest'Aula. Lo dico più da padre

Quasi il 57 per cento. E sapete qual è il dato più drammatico? Quasi la metà di loro ha un giocatore in casa: un padre, un fratello, un amico, una madre, che hanno questo problema. E sapete, di questo

Questa per me è una vergogna! Quanto stiamo facendo con questo decreto è una vergogna e state utilizzando i voti della vostra maggioranza per dare ancora linfa a questo percorso sbagliato. *(Applausi)*.

avete voluto mettere il carico da novanta con questo emendamento. Avete proposto di eliminare totalmente il divieto assoluto di pubblicità indiretta sui giochi che prevedono scommesse e uso di denaro, nonché sul gioco d'azzardo. Per me, questo è stare dalla parte dei lobbisti, non dalla parte dei cittadini. *(Applausi)*. Abbiamo presentato un emendamento per rifinanziare il fondo per il gioco d'azzardo patologico, perché è necessario stare vicino alle nuove generazioni, è importante stare vicino a queste persone, perché sono tutte persone che poi ricadranno sul sistema sanitario del nostro Paese.

in video la vostra presidente Giorgia Meloni diceva che era ben tornata e che farete buon uso di tutte le energie che avete recuperato quest'estate, che siete pronti. Ecco, per me non siete pronti. Anzi, siete pronti a fregarvene degli italiani.

il cosiddetto concordato fiscale perché quanto avete già fatto prima non ha avuto il gettito previsto. Oggi raddoppiate, addirittura con dei costi rilevanti: la relazione tecnica di ieri dimostra che avete dei costi e non dei guadagni. In sostanza, fate in modo che chi fa il furbo e non paga le tasse possa continuare ad evadere, mentre invece a pagare le tasse sono sempre coloro che che hanno un reddito fisso e sono tassati alla fonte. Questa cosa davvero grida vendetta, perché non è accettabile. Addirittura si fa un condono senza pagare pegno:

riequilibrio delle disuguaglianze, la tassazione serve; chi più ha, più dovrebbe pagare. Invece qui ci sono quelli che continuano a fare i furbi e voi li incentivate ad andare in questa direzione. Questo è un dato inaccettabile dal punto di vista del

poteri al commissario, che non c'erano nel decreto-legge iniziale. Sostanzialmente, non solo è stato fatto un decreto il 9 agosto - lo ripeto - ma poi è stato caricato,

Il condono ovviamente viene spacciato da parte vostra come una norma di buonsenso: io evado e il condono è buonsenso. Bisogna essere altruisti nei confronti di chi fa il furbo in questo Paese: si dice, significa lisciare il pelo a quelli che vanno in questa direzione, quindi è un ennesimo incentivo all'evasione, altro che recupero dell'evasione. Non ci piace poi perché avete introdotto il cosiddetto *bonus* Natale,

si è trovata da parte della Commissione la capacità di fare un po' di sintesi in quella direzione). Il cuore di questo decreto-legge - oltre ad essere sbagliato

e una discriminazione per quanto riguarda la questione del reddito, perché si prevede un *bonus*. Anche in tal caso avete criticato i *bonus* e, poi, ne fate uno che discrimina, tra i poveri e non tra i ricchi; come

sul provvedimento, con un suggerimento al Governo; la seconda è una riflessione sul tema di cui si è discusso circa la presenza dei tifosi nella consulta delle società di calcio; infine, farò una riflessione un po' più generale

per chi aveva determinate caratteristiche. Questo rischia di non avere la base su cui fare il calcolo del meno 30 per cento nel periodo Covid. Bisogna quindi trovare una modalità per riempire questo periodo. In tal senso, presenteremo un ordine del giorno (che, ove mai ci fosse la fiducia, decadrebbe e che ripresenteremmo alla Camera) per invitare il Governo a tener conto di questo buco,

relatore mi fa segno di no. Provvederemo con un ordine del giorno e, a questo punto, la soluzione potrà essere operata in via amministrativa, tenuto conto dell'espressione della volontà parlamentare.

Posto il principio, a mio avviso sempre valido, per cui non si legifera sotto emergenza, bisogna fare le leggi ragionandoci bene. Un conto è se c'è un terremoto, ma normalmente bisogna ragionare bene prima di fare una norma. A maggior ragione, mi viene da dire meno male che non siamo intervenuti. La norma La norma non è ancora operativa, però dà un quadro generale e abbiamo tempo per ragionarci bene. Ebbene, come vogliamo intervenire? Ignoriamo completamente il problema, facciamo finta che non esista e mettiamo la polvere sotto il tappeto, oppure rendiamo trasparente il rapporto fra tifoserie e società, come prevede la norma, con una consulta? con quali forme? Come deve essere questa rappresentanza all'interno della consulta? Con quali modalità vengono eletti i rappresentanti all'interno della consulta? Per fortuna abbiamo tempo e, a nostro avviso, è meglio ragionare con calma, ma su questo. L'alternativa di far finta che il problema non esista non mi sembra la migliore. L'ultima questione, abbiamo sentito diversi interventi in tal senso, riguarda i lavori in un periodo particolarmente complicato come questo. nasce già complicato di suo; è stato adottato ai primi di agosto e va da sé che si toglie un mese dei due a disposizione del Parlamento. I lavori su questo decreto-legge hanno stressato al limite al limite il sistema: gli Uffici, le Commissioni e i singoli senatori si sono trovati veramente in difficoltà nel portare a termine il lavoro. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti: gli Uffici, le senatrici e senatori delle Commissioni che comunque hanno dato il massimo per arrivare a chiudere in maniera ordinata il lavoro. Tuttavia, c'è un però. Il Parlamento rischia di fare la fine del vaso di coccio fra i due vasi di ferro. Il Governo Il Governo ha legittimamente l'esigenza di rispondere in tempi rapidi alle istanze che vengono dal Paese, dall'economia e dalla società. Il Quirinale, ancor più correttamente e giustamente, tutela il percorso normativo e la Costituzione. In questo modo, però, i senatori e i deputati vengono sempre più compressi nei loro margini di manovra, come abbiamo visto drammaticamente in questa occasione. Questo è un dato di fatto. Non è una questione del bicameralismo, perfetto sì, perfetto no. Anzi, il bicameralismo perfetto consente di andare al doppio della velocità e quantomeno un ramo del Parlamento riesce a fare un lavoro compiuto (una volta lo fa il Senato, una volta lo fa la Camera). Quindi non è neanche un tema di bicameralismo. Tuttavia - e vengo alla fase propositiva, dopo un'analisi ancorché veloce - dipende anche da noi, dai singoli parlamentari, ritagliarsi e guadagnare spazi di manovra. Mi spiego. Un inciso: ho cinquantasei anni (visto che si parlava di termovalorizzatori, questa la devo dire, perché è uscita nelle discussioni) e cinquantasei sono esattamente gli anni del primo termovalorizzatore di Milano, il primo dei tre. dei tre. Noi abbiamo inserito una norma che prevede, forse, di farne uno in Sicilia, riprendendo una norma che prevede, forse, di farne uno a Roma. Chiusa la parentesi. Due suggerimenti. Il primo le Commissioni, a mio avviso, possono e anzi devono ritagliarsi degli spazi e delle sessioni per compilare dei testi unici. unici. Proprio nelle Commissioni riunite, a proposito dell'agevolazione di 100 euro per le famiglie con redditi più bassi, abbiamo visto quanto è stato complicato fare questo intervento, non per una volontà politica (che è unanime sul tema), ma per la complessità di una materia, quella delle detrazioni familiari, che è complessa, disorganica, confusa, distribuita in tante norme, spesso in contraddizione l'una con l'altra. Ebbene, perché non ritagliarsi un un periodo, una sessione, e non fare un bel testo unico su questa materia? Questo restituirebbe ruolo, dignità e importanza al Senato o alla Camera, a chi volesse fare questo lavoro. E come lo si può fare su questo, lo si può fare su mille altri temi. Il secondo suggerimento è che il Regolamento del Senato prevede la possibilità di fare leggi in tempi molto rapidi con la sede redigente. Facciamone di più. Tantissimi temi non sono potuti entrare in questo, come in altri provvedimenti. Ebbene, facciamo delle leggi velocemente con la sede redigente e invitiamo l'altro ramo del Parlamento a utilizzare le stesse modalità e a copiare lo stesso Regolamento, di modo che si riesca a fare più velocemente il lavoro. La dignità del Parlamento, care colleghe e cari colleghi, dipende soprattutto da ciò che facciamo noi in queste sacre Aule.

il collega presidente Garavaglia, non era difficile prevedere che questo decreto-legge avrebbe avuto un *iter* burrascoso. Peraltro, alcuni dei richiami di metodo che il presidente Garavaglia ha fatto sono pienamente condivisibili anche dalle opposizioni. Quindi la domanda è a chi stia rivolgendo il presidente Garavaglia queste due condivisibili raccomandazioni È stato ricordato che il decreto-legge è stato approvato dal Governo alla vigilia della chiusura delle Camere, comprimendo di fatto i tempi per la discussione parlamentare, recando peraltro un insieme di norme che non ha un filo conduttore unitario. Questo nonostante i continui richiami cui è stata sottoposta la decretazione d'urgenza durante questa stessa legislatura. Nella stesura iniziale del decreto-legge vengono messe insieme discutibili norme di natura fiscale, a partire dal credito d'imposta per gli interventi nel Mezzogiorno, ancora non adeguatamente finanziato (noi l'abbiamo ricordato in molte occasioni), e di proroga di termini normativi; misure di carattere economico con un certo impatto: per esempio il definanziamento del Piano nazionale complementare, cui sono stati sottratti ben 750 milioni di euro, che peraltro sono risorse che in gran parte vanno ai Comuni e agli enti locali. Poi ci sono norme sul controllo pubblico, sul sistema di istruzione, formazione e ricerca, sulle attività culturali, sugli investimenti nel Continente africano (addirittura) e sugli enti territoriali. Su questa varietà di disposizioni, il Governo da una parte e poi la maggioranza dall'altra sono intervenuti *(Brusìo)* non ho capito se la concitazione, Presidente, è conseguente alle mie parole o se sia autonoma, ma proseguo parole o se sia autonoma, ma proseguo - durante i lavori di Commissione, peggiorando, dal nostro punto di vista, il provvedimento e snaturandone ulteriormente la natura di semplice norma tecnica di proroga termini. Non è, fra l'altro, la prima volta che succede: l'abbiamo visto succedere, per esempio, in tempi recenti recenti sul decreto superbonus. Il tempo che ho a disposizione non mi consente di soffermarmi sui diversi colpi di scena che hanno caratterizzato l'*iter* del decreto sui ritardi, sulle sospensioni, in attesa che la maggioranza componesse i propri dissidi e che anche nella giornata di ieri, quindi una giornata festiva, hanno caratterizzato i lavori di Commissione. Faccio questo richiamo di metodo perché prima il presidente Romeo - mi rivolgo a lui ovviamente per suo tramite, Presidente - ha fatto riferimento ad una questione di trasparenza e di metodo. È la stessa questione che noi stiamo ponendo e abbiamo posto anche nella giornata di ieri, quando improvvisamente le Commissioni riunite sono state sospese e la discussione è proseguita altrove. Quindi la questione posta in quest'Aula da alcuni colleghi di maggioranza dovremmo porla noi con forza ai Capigruppo di maggioranza e anche al Governo che è qui presente e che ringrazio. *(Applausi)*. Ma voglio stare al merito e menzionare soltanto due degli emendamenti che avrebbero dovuto e potuto rappresentare non emendamenti ad un decreto *omnibus* di proroga termini fiscali, ma provvedimenti *ad hoc* tali da consentire al Parlamento di svolgere le proprie funzioni e non essere liquidati, come probabilmente accadrà durante questa settimana, con una doppia fiducia al Senato e alla Parlo, *in primis*, dell'intervento del Governo che introduce la pasticciata e discriminatoria norma sul *bonus* tredicesima in busta paga, che peraltro ha escluso dal beneficio i contribuenti con figli nati fuori dal matrimonio. Un provvedimento di quel tipo avrebbe meritato una norma *ad hoc*, il tempo necessario al Parlamento per migliorare un testo che, in questo caso, non è stato assolutamente migliorato dalla discussione in Commissione. Per non parlare del fatto che esiste ormai una sterminata letteratura sui beni collettivi che si è incaricata di dimostrarci quanto, in tempi di incertezza, di inflazione e di risorse scarse, il benessere complessivo dei consumatori - direbbero alcuni economisti - o dei cittadini - diremmo noi - viene incrementato assai di più da interventi pubblici con risorse pubbliche in beni collettivi che nessuno di noi singoli individui è in grado di procurarsi autonomamente sul mercato, piuttosto che in piccole elargizioni *una tantum* destinate a pochi. Nessuno di noi, per esempio, sarebbe mai in grado di acquistare una macchina per fare la risonanza magnetica e sul mercato sanitario del privato una indagine diagnostica di questo tipo costa ben più di 100 euro o 50 euro nel caso il lavoratore sia *part-time* o abbia lavorato soltanto sei mesi durante l'anno. Dovremmo finanziare beni collettivi quando abbiamo poche risorse: sanità pubblica, scuola, istruzione, gli asili nido, che sono stati definanziati da questo Governo nel PNRR, perché con 100 euro le ore che si acquistano sul mercato per una *baby sitter* sono ben poca cosa rispetto all'insieme di risorse che la collettività potrebbe mettere invece su beni che si offrono ai cittadini in maniera collettiva. Il secondo intervento è l'emendamento dei Gruppi di maggioranza - e qui c'è un protagonismo di tutte le forze politiche - che consente di accedere al concordato preventivo biennale con beneficio d'imposta anche a coloro che, negli anni precedenti gli anni del Covid, hanno violato gli obblighi tributari con lo strumento che è stato definito ravvedimento. È un inaccettabile schiaffo ai contribuenti virtuosi, ma non è soltanto questo. Ancora più grave, probabilmente, dal punto di vista della politica fiscale del Governo, è soprattutto la dimostrazione che il concordato preventivo sul quale questo Governo ha fondato la propria riforma fiscale, facendone una bandiera, stenta a decollare per la semplice ragione che il duplice obiettivo di fare cassa e di non disturbare i contribuenti infedeli non può aver successo, perché le due cose non stanno insieme per definizione. Sarebbe meglio che il ministro Giorgetti e il vice ministro Leo prendessero atto di questo fallimento e scegliessero altre strade per finanziare la restante parte della delega fiscale che è rimasta inattuata anche, per esempio, per quanto riguarda il riordino dei tributi alle imprese, di cui sarebbe interessante discutere in quest'Aula, o dei tributi degli enti locali. Si devono invece soltanto alla caparbietà dei colleghi del Partito Democratico (penso al senatore Manca qui presente e al senatore Sensi, che ha parlato prima) le poche note positive del provvedimento: le risorse aggiuntive sul *bonus* psicologico e alcune disposizioni disposizioni sul fronte degli enti territoriali. Purtroppo, signora Presidente, questi pochi segni positivi non sono in grado di cambiare il senso complessivo di un provvedimento che rimane profondamente sbagliato nel metodo e nel merito.

Presidente, onorevoli colleghi, la distanza siderale che, dopo due anni di Governo, divide la nostra maggioranza dalle forze di opposizione, i cosiddetti progressisti dall'uomo della strada, dalla gente che tutti i giorni si alza per andare a lavorare, si misura sui temi che gli altri (quello che fu il campo largo, di cui abbiamo notizie sconfortanti) affrontano in modo ossessivo-compulsivo, come abbiamo sentito dagli interventi che mi hanno preceduto. Tuttavia possiamo dire anche senza persuasione abbiamo fissato bene, nell'album dei ricordi, le profezie degli intellettuali illuminati che, non riuscendo a capacitarsi che gli italiani democraticamente avevano votato una coalizione diversa da quella del loro *main stream*, anticipavano l'avvento delle nuove dieci piaghe d'Egitto: saremmo stati isolati in Europa, il debito sarebbe cresciuto esponenzialmente, l'economia si sarebbe bloccata, la disoccupazione sarebbe esplosa, gli investitori avrebbero sfiduciato i mercati, il PIL sarebbe crollato e non era esclusa l'invasione delle cavallette in monopattino. Purtroppo per loro (e per fortuna per l'Italia), nessuna delle disgrazie si è manifestata, se non quella di un'opposizione abbarbicata su monocordi esternazioni, impegnata a ritrattare gli slanci autonomisti di governatori disattenti alle priorità alluvionali del proprio territorio, ma molto attenti a trovare collocamento in Europa, a rinnegare le riforme sul lavoro votate dal loro partito all'unanimità, a contestare gli accordi con la Libia e la guardia costiera libica senza accorgersi che quegli accordi nell'estate del 2017 erano stati voluti fortemente dal loro Governo e dall'allora ministro Minniti. Poi non stupiamoci se la confusione italiana si riflette nelle votazioni al Parlamento europeo, dove, sulla risoluzione sull'invio delle armi in Ucraina i parlamentari del PD hanno votato per tutto ed il contrario di tutto. Bene ha detto il Presidente del Consiglio, nella prolusione di pochi giorni fa a New York: come politico si hanno due opzioni, essere un *leader* o *follower*, indicare una rotta o no, agire per il bene del proprio popolo o agire solo guidati dai sondaggi. Abbiamo scelto consapevolmente, non senza le note difficoltà ereditate, sulle quali dobbiamo stendere un sudario pietoso, di indicare una rotta e di lavorare giorno dopo giorno per ridare dignità ad una Nazione. Perché quando vediamo la nostra bandiera, noi ne siamo orgogliosi, non ce ne vergogniamo, sentiamo sentiamo l'orgoglio di fare parte di una comunità e siamo pronti a fare la nostra parte per migliorarne le sorti e di farlo velocemente, perché il tempo ce l'hanno già rubato quelli del passato e talvolta dobbiamo occupare il tempo a smentire le gradasse bugie la quale - cito tra le tante - il Governo Meloni avrebbe abolito l'assegno universale. I dati che vi sto leggendo, che non sono stati smentiti, lungi dal rappresentare la lista dei trofei, perché non ci si deve vantare quando si lavora (è un obbligo), è un'analisi sinottica dei risultati ottenuti che hanno consentito più avanti di poter agire anche con il provvedimento che stiamo per licenziare. Quanto emerge è che grazie al Governo Meloni, al dinamismo in politica estera del nostro Presidente del Consiglio, l'Italia ha aumentato i valori delle esportazioni verso moltissimi *partner* commerciali internazionali. Spiccano i dati estremamente positivi dell'*export* verso gli Stati Uniti, Francia, Turchia, Spagna, Cina, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Emirati Arabi Uniti. La nostra Nazione è un fornitore sempre più affidabile e credibile, forte anche del peso che è riuscito a conquistare il marchio *made in Italy* nel mondo. L'Istat ha recentemente pubblicato il rapporto «Conti economici nazionali Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche» negli anni 1995-2023, che rappresenta le stime relative alla revisione generale dei conti economici nazionali, concordate in sede europea, che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti. In particolare, il PIL in volume del 2023 si è attestato a un livello per la prima volta superiore al massimo raggiunto *ante* crisi finanziaria del 2008. Di conseguenza, il *deficit* dello scorso anno risulta inferiore a beneficio della prossima manovra di bilancio del Governo Meloni. Abbiamo dato chiaro il messaggio che lo Stato non avrebbe disturbato chi voleva fare, ma gli sarebbe camminato accanto come un alleato, non come un avversario. Abbiamo detto anche «no» quando dei no andavano detti, perché i soldi dei cittadini non si gettano dalla finestra e quando i soldi non sono spesi adeguatamente, bisogna avere anche il coraggio e la forza di dire no e di non continuare a giustificare, come ho sentito in Commissione misure distruttive - questo era il dato della Commissione - come il superbonus e i banchi a rotelle, con il solo scopo di lavarsi la coscienza sporca dai danni fatti quando si era al Governo. Nel 2023 l'Italia cresce più del doppio della media UE e dell'Eurozona. L'Italia cresce del + 0,9, con una media europea del + 0,4. Per quest'anno la Commissione europea prevede che l'Italia cresca dello 0,9, una previsione più alta di quella prevista per l'Eurozona, di quella prevista per la Germania, di quella prevista per il vostro esempio francese. francese. Stiamo andando meglio degli altri, anche se sarebbe stupido rallegrarsene, perché la debolezza - come si ricorda correttamente - di alcune economie europee frena anche la nostra crescita, soprattutto dell'industria tedesca, che chiaramente, per molte delle nostre imprese, è uno sbocco fondamentale. La borsa ha superato il livello pre-crisi finanziaria del 2008, sta facendo registrare la migliore *performance* in Europa e tra le migliori *performance* nel mondo. Lo *spread* è a un livello di circa 100 punti base inferiore rispetto a quello dell'ottobre 2022. Poi, ovviamente, c'è il mercato del lavoro: i dati Istat di luglio ci dicono che abbiamo superato per la prima volta i 24 milioni di lavoratori. Mai così tanti italiani avevano lavorato dall'Unità d'Italia a oggi. Il tasso di occupazione generale ha raggiunto il 62,3 per cento, quello di occupazione femminile il 53,6, superando per la prima volta il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici. Anche questo è qualcosa su cui il Governo ha lavorato, concentrando le risorse particolarmente sulle mamme lavoratrici, come la grande sfida dell'occupazione femminile in Italia e delle donne. Lo dovevamo alle nostre nonne, che questa Patria, nel Novecento delle due Guerre mondiali, l'hanno costruita e fatta forte. Tendenza opposta è il tasso di disoccupazione che scende a luglio al 6,5 per cento, il più basso dal 2008. *(Applausi)*. Dall'ottobre del 2022 si contano circa 750.000 occupati in più: 408.000 dei quali sono donne. È un'occupazione di qualità, visto che salgono gli occupati a tempo indeterminato. Potrei continuare, ma non voglio distrarmi da quello che è l'obiettivo: creare le basi per sviluppare le altezze. Questo lo si fa anche con provvedimenti come questo, dove - come dicevo prima si cammina a fianco ai cittadini, ai nostri sindaci, alle tante attività commerciali, industriali ed associative che creano esse stesse i risultati citati sopra. Abbiamo affrontato la ZES unica, il lavoro sportivo, i grandi eventi culturali come quello nella mia Gorizia che, insieme a Nova Gorica, sarà nel 2025 Capitale europea della cultura. Abbiamo sostenuto tutti quei territori, vittime di troppi anni di chiacchiericcio e incuria, liberando le risorse dei fondi di emergenza destinati. Signor Presidente, stiamo aggiungendo anche oggi un altro tassello al grande obiettivo che ci siamo prefissati due anni fa, alla promessa cardine: rimettere al centro dell'azione politica la grande energia dei nostri cittadini, per far tornare la nostra grande Italia grande nel mondo.

onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: - all'articolo 2-*quater* (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";

"Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante misure di carattere fiscale ed economico, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5a e 6a con le modifiche richieste dalla 5a Commissione. Domani, alle ore 10, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama. Sarà discusso inoltre, dalla sede redigente, il disegno di legge sull'insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'educazione civica. La discussione del disegno di legge sulle manifestazioni di rievocazione storica inizierà mercoledì 2 ottobre. Per il *question time* di giovedì 3 ottobre è prevista la presenza dei Ministri degli affari esteri, delle imprese e per le riforme istituzionali. Il Parlamento in seduta comune potrebbe essere convocato martedì 8 ottobre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. La discussione del Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine, già deferito alla Commissione bilancio, inizierà mercoledì 9 ottobre. Di conseguenza, la giornata di martedì 8 sarà riservata ai lavori delle Commissioni. La settimana dal 21 al 25 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Mercoledì 2 ottobre la seduta sarà sospesa dalle ore 13 alle ore 15,30.